Grazie

erano presenti. Per un problema puramente tecnico non siamo ancora riusciti a definire una modifica del calendario che renda possibile il rispetto di questo impegno. Quindi affido a lei e all'Assemblea tale esigenza, sperando di trovare una soluzione rapida, magari con una convocazione lampo della Conferenza dei Capigruppo che modifichi il calendario.

Martedì scorso abbiamo concluso il dibattuto su un tema delicato ed importante per l'opinione pubblica come quello sulla gestione delle banche e lo abbiamo fatto in un clima estremamente positivo,

Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia si associa alla richiesta, perché martedì si possa arrivare al termine della discussione delle mozioni sulle banche, che riteniamo sicuramente importante. Del resto, quando è stata interrotta la discussione era abbastanza palese che l'intendimento

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, vorrei approfittare dell'occasione di questa replica per fornire dei chiarimenti, qualora vi fossero ancora dei dubbi, perché mi pare che ieri, nell'ambito della discussione generale qualche collega,

prevede che le Province e i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i Consigli regionali, sia approvato con legge della Repubblica.

dalla Regione Veneto e l'annessione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale. Non vi è, pertanto, la necessità di una legge costituzionale. Le disposizioni richiamate si riferiscono a tutte le Regioni, senza deroghe alla procedura, qualora una delle Regioni interessate, come nel caso di specie, sia dotata di uno Statuto approvato con legge costituzionale.

dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle D'Aosta. Ricordo altresì che tale necessità è esclusa dall'articolo 46 della legge n. 352 del maggio 1970.

che in maniera così approfondita e articolata hanno avuto modo di dibattere sull'argomento, e in particolare l'allora presidente della Commissione Anna Finocchiaro e l'attuale presidente Salvo Torrisi,

è iniziato nell'ottobre del 2013 e vorrei anche ricordare in maniera molto opportuna - mi sta particolarmente a cuore - che il *referendum* popolare che la comunità di Sappada ha svolto nel 2008 ha

procedura indicata: continuità geografica, omogeneità economica e sociale, vicinanza storico‑culturale del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Non è una questione solamente economica, ma molto più complessa; ha profonde radici storico-culturali e anche linguistiche.

attende questo voto da parte del Parlamento. Oggi arriviamo a poter dare finalmente una risposta, dopo molti anni di attesa, alle esigenze di un'intera popolazione. Sappiamo che questo è un voto molto significativo; la condivisione in Commissione è stata è stata ampia e mi auguro che in maniera molto veloce si possa procedere anche in questa Assemblea, proprio a significare un passaggio atteso e fondamentale che dà risposta

Lo dico al collega Sonego, perché il tema dell'etnia, in termini antropologici, nulla ha a che fare con la vicenda di Sappada. Casomai c'è un tema di comunanza di costumi, di socialità di socialità condivisa dentro lo Stato, infraconfine e non extraconfine. Quindi non si tratta di un'affermazione etnica, ma di un ricongiungimento di comunità, all'interno di una diversa entità amministrativa locale.

non nego la contestualità, ma di certo le ragioni hanno più a che fare con la storia, che non con l'attuale contesto amministrativo e istituzionale.

il tema va affrontato con rigore e senza rinunciare alle responsabilità, ma senza attenuare la responsabilità del non fatto. Sappada è storicamente carnica: è stato detto in diversi interventi e ciò è testimoniato, oltretutto, dalla continua appartenenza alla diocesi di Udine. La rottura è avvenuta a metà dell'Ottocento, a causa di un dominio esterno

alla più vasta comunità carnica. Appunto per questo la rilevanza non è la specialità, ma la comunità.

raro, di una condizione davvero specifica e particolare, puntuale e non estensibile ad altre situazioni. Vorrei infine dire, in ordine al tema dello strumento che in fatto di costituzionalità il Servizio studi del Senato è stato chiaro, affermando che: «la procedura descritta si applica anche quando, come nel caso in esame, si prevede il distacco di un ente locale da una Regione a statuto ordinario (nel caso di specie il Veneto) e l'aggregazione ad una Regione a statuto speciale (nel caso di specie il Friuli-Venezia Giulia). La procedura prevista all'articolo 132, secondo comma, non distingue infatti fra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale (i cui confini sono individuati dagli statuti approvati con legge

disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni», al secondo comma non fa alcun riferimento a leggi di rango costituzionale e dice semplicemente che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica (...)». Quindi non è in alcun modo richiamata la necessità di una norma di rango costituzionale per il passaggio del Comune di Sappada dalla Regione Veneto alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Per queste ragioni il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di legge e anticipo già

riguarda la copertura finanziaria della presente proposta, la decorrenza a partire dall'anno 2017, perché ovviamente il testo è stato licenziato dalla Commissione l'anno scorso e quindi occorreva aggiornare

la voce di una popolazione che in questi mesi ha scelto di non urlare e di portare avanti le proprie istanze con esemplare determinazione e innata dignità. Mi chiedo e vi chiedo, cari colleghi, può la politica permettersi di non ascoltare? O peggio, come accaduto in questi mesi per Sappada e come accade da troppi anni per tutti gli altri Comuni referendari del bellunese (e non solo, ma dell'intera nostra nazione), può far finta di non sentire? Oggi, colleghi, è una giornata importante, lo dicevo ieri e lo ribadisco in conclusione di questo mio intervento; penso lo sia anche in termini di responsabilità e di riflessione sul ruolo della politica e del Parlamento. È quindi doveroso da parte mia anche ringraziare i membri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio per aver compreso le motivazioni del disegno di legge in esame e dei cittadini di Sappada. Oltre alla

Il perché di questo atteggiamento è noto, direi tristemente caratterizzante e insieme distante dai doveri, le funzioni e i compiti che è chiamato a svolgere chi ha il privilegio di sedere tra questi banchi. Oggi Sappada volta pagina e chiedo scusa ai sappadini per i ritardi che hanno dovuto subire a causa di altre persone, di altri colleghi, o della politica in genere che non ha voluto ascoltare le loro richieste. Chiedo scusa a loro e ai cittadini di tutti i Comuni referendari che da troppo tempo attendono risposte dovute e non più rinviabili ed ai quali esprimo piena solidarietà.

che la politica è vicina ai cittadini.

in favore della popolazione sappadina che da dieci lunghi anni attende che il via libera del Parlamento dia corso ad una istanza che ha trovato ragione in un *referendum* e che, in seguito, è stata avallata dai Consigli regionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

che, come tante altre domande pervenute da diverse località italiane, è rimasta purtroppo giacente per anni, contravvenendo così ad una precisa volontà democraticamente espressa da una comunità intera nell'ormai lontano 2008. Siamo chiamati, senza ulteriori indugi e senza esitazioni di sorta, a dare il via libera al ricongiungimento di una comunità, quella sappadina, che geograficamente, storicamente e culturalmente è legata alla Carnia. La norma in esame, che io stesso promossi da cofirmatario nel 2013, è in sostanza un atto dovuto anche in forza del principio internazionalmente riconosciuto dell'autodeterminazione dei popoli

e nella volontà di non imporre altri ostacoli a questo diritto, ci consente di approvare questa norma senza le formalità e le maggioranze stabilite, invece, per una legge di rango costituzionale. L'occasione rappresentata da questa votazione ci permette però di portare alla luce anche un'altra grande problematica che affligge il comprensorio delle Dolomiti venete ed in particolare tutto il Cadore. la richiesta forte e chiara giunta da Sappada, oltre a trovare le proprie radici nella storia, nella lingua, nella tradizione di una comunità che ha origini germanofone e tratti comuni con le vicine località della Carnia, è motivata, inevitabilmente, anche da un fattore economico. Non sfugge, infatti, che tutto il Cadore, così come altre zone montane e pedemontane del Veneto confinanti con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, soffrono oggi di un *gap* enorme nei confronti delle vicine località trentine e friulane che possono godere di tutti gli innegabili benefici provenienti dalla amministrazione autonoma regionale. La disparità tra Regioni ordinarie e Regioni autonome in questi territori montani del Veneto, e non solo lì, è estremamente evidente e viene vissuta ogni giorno sulla pelle dei cittadini. Servizi, infrastrutture, promozione turistica, interventi di sostegno per lo sviluppo di nuove attività ricettive e commerciali sono nettamente diversi tra Veneto da una parte e Trentino e Friuli dall'altra. Una situazione questa che, negli anni, ha provocato un netto arricchimento del Sudtirolo, lo sviluppo turistico della Carnia e, allo stesso tempo, un progressivo impoverimento delle attigue località bellunesi. È indubbio, infatti, che la realtà delle Regioni autonome ha favorito lo sviluppo dei territori che hanno potuto godere di tutti i benefici costituzionalmente garantiti per queste zone; così non è stato per il bellunese, ma anche per parti del vicentino e del feltrino che soffrono una situazione economica di minor benessere rispetto ad altri comuni confinanti, ma appartenenti a Regioni diverse. Una condizione che non ha soltanto risvolti economici ma anche sociali e che si traduce inevitabilmente nel fenomeno dell'abbandono delle comunità montane venete da parte dei giovani costretti a recarsi altrove alla ricerca di un lavoro e della possibilità di condurre una vita dignitosa. Dunque la volontà espressa dalla comunità di Sappada, che ha delle fondate ragioni per chiedere di essere aggregata alla provincia di Udine, deve giungere in quest'Aula anche come una richiesta di maggiore attenzione da parte del Governo, dell'amministrazione e - non ultimo - del legislatore nei riguardi di interi territori costretti oggi a fare i conti con una limitata disponibilità di strumenti per far fronte alla sempre più competitive offerte turistiche e sociali delle zone limitrofe. Una problematica che non è risolvibile con una serie infinita di distaccamenti dal Veneto e aggregazioni alle Regioni confinanti, ma che richiede, anche nel rispetto dell'articolo 9 della nostra Costituzione, l'adozione di una politica di valorizzazione e sostegno alle aree montane e pedemontane che custodiscono una parte rilevante del patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro territorio. Diversamente rischieremo nei prossimi anni di dover ridisegnare in maniera marcata i confini non solo di queste Regioni ma anche di altre che in Italia si trovano a vivere la stessa condizione di svantaggio. Auspicando che le misure necessarie a sostenere le aree montane meno sviluppate possano essere elaborate ed adottate presto e bene e nuove politiche di sviluppo siano concepite per questo e per moltissimi altri territori più svantaggiati, ribadisco l'appoggio del Gruppo Federazione della Liberta alla legittima richiesta avanzata da questa comunità di nostri connazionali che per cultura, sentimento e tradizione gravita sulla provincia di Udine, di cui peraltro è stata parte integrante fino al 1852, e che già da molto tempo, troppo, attende una risposta in questo senso per riprendere a vivere e sperare in una condizione che essa stessa considera migliore.

gli argomenti e la problematicità emersi nel corso della discussione su questo disegno di legge, sia in Commissione che in Aula, ci portano a guardare con attenzione e in qualche modo con preoccupazione a procedure finalizzate alla variazione dei confini regionali. Preoccupazione che è stata colta in interventi di diversi colleghi e che il nostro Gruppo condivide. Oggi però si tratta di esprimere il proprio orientamento su un caso concreto ed è a questo che dobbiamo guardare per esprimere il nostro orientamento e il nostro voto. Il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione al Friuli-Venezia Giulia avviene a fronte di una espressione di volontà in questo senso quasi plebiscitaria

Avviene inoltre con il parere favorevole dei Consigli delle due Regioni coinvolte e soprattutto avviene sulla base di solide ragioni storiche, culturali e linguistiche a favore della ricostituzione di una comunità che, pur divisa dal punto di vista geografico, non ha mai visto venire meno i solidi legami che la tengono unita. Nel merito, pertanto, il disegno di legge va nella direzione giusta. Aggiungo che anche sul piano procedurale non emergono problemi di sorta e, anzi, appare pienamente rispettata la normativa vigente a partire dall'articolo 132, secondo comma della Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo aggiungo, con riferimento alla circostanza che stiamo per sancire il passaggio da una Regione a statuto ordinario ad una Regione a Statuto speciale, che la procedura prevista in Costituzione non prevede alcuna distinzione ed è applicabile al passaggio da una Regione a un'altra a prescindere dal fatto che si tratti di Regioni a statuto ordinario o di Regioni a Statuto speciale. Anche il Sottosegretario, che ha espresso il parere del Governo, poco fa ha sottolineato questa circostanza. Per queste ragioni, condividendo nel merito il disegno di legge, che ha alle spalle un *referendum* e il parere delle due Regioni coinvolte, a nome del Gruppo Articolo 1 - MDP, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi dal Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comune di Sappada finalmente passa dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. I cittadini di Sappada si sentono friulani, da sempre vicini a quel territorio; una vicinanza che si esprime non solo in termini di contiguità geografica, ma anche per struttura economica e vicinanza storico-culturale. Il *referendum* è stato stravinto dal sì con il 95 per cento dei voti e a nove anni da questo evidente risultato è chiaro e necessario che i cittadini debbano avere una risposta definitiva. Sappada, fino al 1852, faceva parte della provincia di Udine e i legami socio-culturali sono certamente rimasti, compreso il dialetto delle zone. Al di là delle ragioni economico-culturali, sono favorevole a questo distaccamento perché la volontà popolare deve prevalere, perché così specifica la nostra Costituzione, al di là di qualsiasi calcolo o schieramento politico. Non a caso i diritti popolari esercitabili soprattutto attraverso iniziativa legislativa e *referendum* rappresentano una prerogativa non negoziabile. Il mancato rispetto dell'espressione della maggioranza dei votanti sarebbe devastante in una democrazia del nostro tipo e rischierebbe di creare un solco sempre più profondo fra cittadini e Stato Stato e davvero non ce lo possiamo permettere. Lo scopo è quello di creare una classe politica capace di rispettare la volontà popolare, anche e soprattutto quando si manifesta con orientamenti differenti dai desideri di parte, per colmare sempre più il *deficit* di rappresentanza vissuto da molti cittadini. Signor Presidente, per tutti questi motivi, dichiaro il mio voto favorevole e quello del mio Gruppo Grandi Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprime, nel merito, una posizione favorevole: noi pensiamo che il voto referendario e la volontà dei cittadini di Sappada debbano essere rispettati. Vi sono, inoltre, i pareri positivi delle Regioni interessate.

Esprimiamo, invece, una perplessità in merito allo strumento utilizzato, cioè la legge ordinaria. Noi da sempre - e non solo noi, ma anche grande parte della dottrina che per modificare il territorio di una Regione a statuto speciale serva una legge costituzionale. Ciò per il semplice motivo che il territorio della Regione a Statuto speciale è disciplinato dallo statuto stesso, cioè da una norma

se si consentisse con legge ordinaria questo passaggio, verrebbe totalmente snaturata la natura della Regione a Statuto speciale, la composizione linguistica bellunesi venissero aggregati alla Provincia autonoma di Bolzano, anche i rapporti tra i vari gruppi linguistici. Pertanto siamo dell'avviso che bisognerebbe agire con una legge costituzionale. Per questa ragione, anche noi, proponendo il passaggio dei tre Comuni di Cortina d'Ampezzo,

la Corte consente la legge ordinaria come strumento e non lo impone. Sarebbe quindi più opportuno procedere in questo modo, anche per evitare precedenti negativi, poco rispettosi delle autonomie speciali. speciali. All'interno del nostro Gruppo non abbiamo tutti una posizione unanime al riguardo. Come ho detto, nel merito condividiamo il passaggio del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ma con uno strumento che a noi non sembra quello più appropriato. Per questo motivo una parte del nostro Gruppo voterà a favore e un'altra parte si asterrà. [DALLA Signor Presidente, anticipo che il mio Gruppo voterà «sì», però devo dire con forza che sia in Parlamento sia nella Regione Veneto c'è una grande ipocrisia su quello che stiamo dicendo e facendo: questa è la mia opinione.

sì a sedici Comuni, se vogliamo essere coerenti con quello che stiamo dicendo. La stessa cosa devono fare il Consiglio regionale del Veneto, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e i Consigli provinciali del Trentino-Alto Adige. Adesso il collega Zeller ha detto che è disponibile a ricevere Cortina, come a dire: dateci l'oro che a noi fa bene, ma il resto non lo vogliamo. È facile ragionare in questo modo. Perché questi trentuno La realtà vera è che anche qui c'è una grande mistificazione: si parla di cultura, di tante cose, di storia, di etnie. La banalità è una sola: i cittadini di quei Comuni al confine vedono la differenza dei trasferimenti dello Stato alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Non prendiamoci in giro. In tutti i Comuni di confine ci sono storie, culture diverse e quant'altro. Quindi dobbiamo dire pane al pane e vino al vino. Lo Stato per sopperire a questa difficoltà ha varato diverse leggi sulle aree di confine; ricordiamo,

Grazie

che stiamo aprendo una strada che sottovalutiamo e a cui, forse, diamo la risposta sbagliata.

di un'*enclave* germanofona e di una comunità che ha affinità culturali e di tradizioni storiche

grazie a tutta

solamente oggi, undici anni dopo l'avvio dell'*iter*, è emblematico del baratro che separa questi Palazzi dai territori e della scarsa attenzione - voglio essere cortese - che la maggioranza rivolge alla legittima volontà dei cittadini e delle amministrazioni locali. Undici anni sono passati e mai sono comparse difficoltà o elementi ostativi, eppure i sappadini ancora sono sospesi in attesa che vengano riconosciuti la loro volontà e i loro diritti. Non ci si stupisca, poi, se alle amministrative il partito di governo continua a prendere bocciature sonore ed emblematiche. Penso a Genova e Pistoia, ma anche a Carrara, Fabriano e Guidonia, dove è stato scelto il Movimento 5 Stelle. E a poco giova presentarsi, più o meno mascherati, dietro il paravento di altre liste civiche, perché se è questo il modo con cui le maggioranze di governo occupano il Parlamento, la loro distanza dai cittadini è ormai siderale. Passatemi un'amara battuta: il vero distacco non è quello del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, ma quello tra PD e grazie a tutta per il passaggio di Sappada alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. La votazione si è tenuta nelle giornate del 9 e 10 marzo 2008: l'affluenza è stata pari al 75,3 per cento e i sì hanno vinto con il 95 per cento dei voti. Il 18 marzo 2009 il Consiglio provinciale di Udine ha approvato l'ordine del giorno per il passaggio di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sia il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il 23 novembre 2010, che quello del Veneto, il 28 giugno 2012, hanno espresso il proprio parere favorevole. L'8 gennaio 2014 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso anch'essa parere favorevole. Poi, malgrado fosse un disegno di legge semplice e condiviso, che si sarebbe potuto licenziare in poche ore, alla volontà popolare non si è mai dato spazio nel calendario della 1ª Commissione, occupato com'era dalle "deforme" del PD renziano. Mi riferisco alla sciagurata legge Delrio, che ha finto di abolire le Province, ma le ha solo dissestate e sottratte al voto popolare, e alla finta abolizione del finanziamento ai partiti, riformulato sotto mentite spoglie, per finire poi con una legge elettorale incostituzionale e valida solo per una Camera, di cui vediamo adesso gli effetti, perché tanto poi avrebbero riparato con la riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione è stata cioè degradata a sanatoria di una legge ordinaria. trattava di una "deforma" di cui l'Italia avesse necessità, perché altre erano le urgenze, ma serviva al PD per blindarsi il potere. Queste sono le logiche. I tempi in Commissione sono sempre stati decisi dal Partito Democratico, forzando quando servivano annunci propagandastici e rallentando quando dava loro fastidio. Così sono stati congelati la legge sul lobbismo, quella che tutela chi denuncia la corruzione (la cosiddetta *whistleblower*) e molti altri provvedimenti come questo disegno di legge, mentre sono passati avanti provvedimenti che onestamente, colleghi, non potete definire prioritari. Ci sono voluti oltre due anni perché questo provvedimento venisse messo in calendario e, a quel punto, è bastato verificare che la richiesta rispettava ampiamente i requisiti di continuità geografica, omogeneità economica e sociale e vicinanza storico-culturale del Comune di Sappada alla Regione di destinazione, un passaggio pressoché scontato e rapidissimo. Poi, di nuovo, il nulla. Malgrado reiterate proteste e denunce delle istituzioni locali, oggi che, siamo a settembre 2017 ed è passato un altro anno e mezzo, ci avviciniamo al termine della legislatura e ancora manca il passaggio alla Camera. Perché? Dobbiamo forse pensare che ci sia una sorta di allergia della maggioranza di Governo - e del Partito Democratico, in particolare - a recepire la volontà popolare? I fatti lo indicano. Pensate al fastidio per la consultazione popolare su una possibile maggiore autonomia per Veneto e Lombardia: Governo e PD hanno avuto il coraggio di dire che sono soldi sprecati. Sarebbe uno spreco chiedere ai cittadini cosa vogliono veramente? Per voi magari sì, ma ricordo che questo presunto spreco l'ha voluto il Governo, negando l'*election day* che avrebbe consentito, quello sì, di risparmiare 14 milioni di euro pubblici. La refrattarietà del PD alla volontà popolare, però, ha origini lontane: lo abbiamo visto con il tradimento dell'esito del *referendum* sull'acqua pubblica del 2011, prima trattato con sufficienza, poi, all'ultimo momento, condiviso, sull'onda di milioni di firme, e poi definitivamente tradito in questa legislatura con la legge Madia. Abbiamo visto com'è stato vilipeso il *referendum* contro le trivellazioni nel 2016: i cittadini hanno raccolto milioni di firme per sei *referendum*, il Governo si è spaventato e che ha *In extremis*, ha cambiato la legge, falciandone cinque; sul superstite è calato poi il silenzio di Stato della nuova RAI voluta dal PD, durante la campagna referendaria. Stesso giochino con il *referendum* sul lavoro, con l'aggiunta di una beffa atroce sui *voucher*: ancora una volta, i cittadini hanno raccolto milioni di firme, ma il Governo ha cambiato la legge, per evitare un *referendum* che sarebbe stato una valanga per il Partito Democratico poi, scampato il pericolo e vilipesi i cittadini, sostanzialmente ha reintrodotto i *voucher*, con caratteristiche, per alcuni versi, assolutamente identiche. Ci rendiamo conto dell'affronto alla democrazia? Che importanza può avere dunque, signor Presidente, per questa maggioranza, che tradisce un'intera Nazione, la richiesta di una comunità locale? In questi mesi, sia in Conferenza dei Capigruppo, sia in il Movimento 5 Stelle ha più volte chiesto la calendarizzazione del provvedimento in esame, trovando un muro di gomma di voti contrari e di rinvii ad opera della maggioranza. Oggi, che magari paga, più a ridosso delle elezioni politiche, si intravede una lucina in fondo al tunnel in cui era piombato questo provvedimento. lo ripeto, manca il passaggio alla Camera e qui voglio ribadire qualche concetto d'assoluta importanza. Il primo è che il Movimento cinque Stelle è, per i suoi principi, favorevole a tutti gli strumenti di democrazia diretta, *in primis* il *referendum*, che ne è la massima espressione. secondo è che il Movimento Cinque Stelle si oppone e si opporrà strenuamente al soffocamento dei territori che si ribellano. Dalla Tor, perché va difesa la volontà popolare dei Comuni Veneti, quando è legittima e basata su un diritto. Non possiamo addurre motivazioni oblique che esulano dal merito specifico e dalla valutazione attenta della legittimità della richiesta. Ogni altra comunità che affermi i principi di autodeterminazione nel rispetto della Costituzione della Repubblica va rispettata. Noi abbiamo dimostrato questo rispetto con la battaglia in difesa della Costituzione e delle autonomie locali, vinta il 4 dicembre 2016. Lo dimostriamo oggi, nel rispetto di quanto enunciato dall'articolo 132 della Costituzione, esprimendo, ovviamente, voto favorevole al disegno di legge facoltà. PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Il disegno di legge ordinaria alla nostra attenzione è costituito da un unico articolo che disciplina la procedura per il distacco del Comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia conformemente al procedimento di cui all'articolo 132, comma 2, della Costituzione. Ovviamente la previsione contenuta nel testo in esame tiene conto della decisione espressa con il *referendum* consultivo del 9 e 10 marzo del 2008 della comunità di Sappada. Essa, superato il *quorum* previsto dalla legge n. 352 del 1970, con il 95 per cento dei voti a favore, ha scelto di aderire alla Regione con cui confina, lasciando la Regione Veneto cui attualmente appartiene. Del resto, le due Regioni coinvolte dalla variazione territoriale hanno manifestato il proprio parere favorevole, come richiesto dalla norma costituzionale, offrendo in questo modo al Parlamento un ulteriore elemento, sia pure non vincolante, così come in senso favorevole si sono pronunciate la Provincia di Belluno e quella di Udine. Sappada, com'è stato detto, è un piccolo Comune (1.300 abitanti) a ridosso dell'omonima cima dolomitica, sulle Alpi Carniche, attraversato dal fiume Piave. La storia di Sappada parte dal X secolo ed è prevalentemente legata alla Provincia di Udine, che lascia nel 1852, per passare a quella di Belluno. Nel paese, che è una località a forte vocazione turistica invernale ed estiva, dotata di un patrimonio ambientale straordinario, sono presenti tre differenti musei (etnografico, della civiltà contadina e della Grande Guerra) sinonimo di una vivace varietà di iniziative culturali ed artistiche fortemente radicate nella tradizione locale. Nella valorizzazione della propria tradizione e della propria cultura e nel riconoscimento di Sappada come isola linguistica germanofona è stato elaborato anche un vocabolario del del dialetto sappadino, nato dall'esigenza di creare uno strumento alla portata di chiunque voglia consultarlo. Insomma, ci troviamo di fronte a una realtà attiva che, considerata la propria origine e la propria stona civile e religiosa, si riconosce certamente di più nella realtà friulana che in quella veneta. Dunque, un insieme di singolari caratteristiche, le quali, a un primo e superficiale approccio, potrebbero essere sufficienti a motivare il distacco. Signor Presidente, è necessario però approfondire ulteriormente la questione: la richiesta degli abitanti di Sappada riporta al disagio economico e sociale vissuto quotidianamente dai territori ordinari adiacenti ad aree di Regioni a ordinamento differenziato. La richiesta di Sappada riporta all'esigenza concreta di un territorio montano di ammodernare l'offerta turistica nella parte impiantistica e nella parte ricettiva, e risponde alle necessità di chi opera, di chi intraprende, di chi fornisce servizi e di chi ne fruisce. Riguarda cioè la vita quotidiana di cittadini, imprese ed enti. Risponde inoltre all'esigenza di disporre di adeguati strumenti amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo del territorio. Non c'è dubbio che una delle motivazioni che hanno sostenuto il largo successo del *referendum* tra la popolazione sta nell'esigenza di poter guardare verso un futuro caratterizzato da condizioni economiche, amministrative e legislative più favorevoli allo sviluppo. In altre parole, i tentativi di migrazione verso le Regioni a Statuto speciale da parte dei territori ordinari sono determinati da forti squilibri esistenti che si ripercuotono, particolarmente in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole, sulle piccole realtà locali, in particolare su famiglie ed imprese, determinando spopolamento ed impoverimento economico-sociale. Non solo i Comuni confinanti con il Friuli come Sappada, ma numerosi altri della Provincia di Belluno si sono pronunciati a favore del passaggio ad altra Regione

e ben 35 Comuni che confinano, ad Ovest, con il Trentino-Alto Adige. In assenza di azioni incisive che affrontino la condizione cui ho fatto cenno, ci si troverà di fronte ad un vero e proprio effetto domino devastante per la Provincia di Belluno e ingovernabile, nel caso dell'altra parte del territorio veneto, motivato da anacronistici privilegi e garanzie che peraltro la riforma costituzionale bocciata il 4 dicembre non aveva neppure - colpevolmente - lontanamente affrontato, svelando un'azione politica del Partito Democratico incapace di dare le dovute risposte di equità e di parità di possibilità competitive alle popolazioni interessate, insieme all'incapacità di affrontare il disegno di un nuovo ed efficiente governo del territorio, con ciò esprimendo, a mio avviso, l'arroganza politica di questa posizione e la mancanza di volontà di ascoltare ed accompagnare i territori. D'altronde, proprio le resistenze manifestate in più occasioni verso la calendarizzazione di questo provvedimento sono l'ulteriore prova della insensibilità verso il problema. Le risposte attese dalle popolazioni interessate riguardano dunque la relazione esistente tra territori cosiddetti ordinari e territori a Statuto speciale, con tutto il carico di disparità di trattamento che questo porta con sé. Proprio per questo, ed al fine di contribuire alla ricerca di soluzioni praticabili, avevo presentato ed avevo richiesto più volte la calendarizzazione del disegno di legge n. 2279 condiviso dall'Associazione dei Comuni di confine, concernente azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, riprendendo il modello dei Fondi di confine riconosciuti ai territori veneti e lombardi confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e noti come fondi Calderoli-Brancher, migliorando, se possibile, le modalità di erogazione soprattutto in merito al profilo strategico attribuito a tali fondi. Fosse stato avviato un serio esame, presupposto di provvedimenti adeguati, ora, con elevata probabilità, non ci troveremmo qui a trattare l'argomento all'ordine del giorno. Neppure le ordinarie azioni consentite agli enti locali e territoriali possono venire in aiuto, atteso che gli ultimi Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno ridotto all'impotenza i Comuni, hanno eliminato la concreta possibilità di programmi territoriali adeguati da parte delle Regioni a statuto ordinario, hanno eliminato l'operatività delle Province quale effettivo strumento di coordinamento e programmazione attraverso l'attuazione della legge Delrio, portandole letteralmente al disastro operativo e finanziario. Sono certo che il *referendum* consultivo che si celebrerà in Veneto e Lombardia il prossimo 22 ottobre contribuirà a chiarire a tutti che è necessario attribuire ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, procedendo ad un indispensabile riequilibrio del sistema amministrativo del nostro Paese

permettere ai sappadini di intraprendere questa nuova strada, auspicando allo stesso tempo che Parlamento e Governo rispondano con urgenza ed in modo organico alle pesanti questioni che la decisione di oggi lascia irrisolte dietro di sé. Con ciò, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. come ripetutamente richiamato anche da molti colleghi che mi hanno preceduto, quest'oggi finalmente il Senato è chiamato ad approvare un disegno di legge che - dobbiamo ammetterlo - arriva all'esame di questa Assemblea con qualche colpevole ritardo. Infatti, la norma che, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, dispone il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia nasce come risposta, eufemisticamente poco tempestiva, all'iniziativa assunta da quel territorio addirittura dieci anni fa, quando il Consiglio comunale formulava la richiesta di *referendum* popolare consultivo per permettere ai cittadini di esprimere la loro opinione in merito. Ebbene, come sappiamo, la volontà dei sappadini è stata chiara: la votazione si è tenuta il 9 e 10 marzo 2008 e, su un totale di 1.199 aventi diritto, come è stato ricordato, si sono recati alle urne 903 elettori, il 75 per cento, e di questi ben 860 si sono pronunciati per il sì: il 95 per cento. Aggiungo, allora, a quanto emerso in questo dibattito due brevissime considerazioni e una riflessione legata all'attualità di quanto succede in queste ore in Europa. Chiunque conosca la realtà di quel territorio, sa che le ragioni dei sappadini sono, dal punto di vista storico, assolutamente fondate. Pur facendo parte da più di centocinquant'anni della Provincia di Belluno, Sappada mantiene un'originaria identità culturale e linguistica germanofona, che affonda le sue radici probabilmente nell'insediamento di un nucleo di famiglie austriache nell'XI secolo. Da quel momento Sappada appartenne alla gastaldia della Carnia (incorporata nel 1420, insieme a tutti i territori del patriarcato, nel dominio della Repubblica di Venezia), e, appena dopo l'alternarsi delle dominazioni francese e austriaca, venne staccata dalla Carnia, quindi dal Friuli, nel marzo del 1852, quando dalla Provincia di Udine passa a quella di Belluno (già allora tra le proteste dei suoi abitanti). Va ricordato inoltre che, durante la Seconda guerra mondiale, il paese fece parte della Repubblica libera della Carnia e che per la giurisdizione ecclesiastica è rimasta, senza soluzione di continuità, legata alla diocesi di Udine, erede del soppresso patriarcato di Aquileia. Dal punto di vista culturale, quindi, non vi è dubbio che Sappada presenti fortissime affinità con le vicine comunità carniche, con cui condivide da sempre, oltre che il profilo delle comuni montagne, cultura, valori, territorio, destino e disagi, e che il *referendum* di dieci anni fa rappresenti una forte e legittima richiesta di autogoverno e di amministrazione alpina capaci di coinvolgere e rilanciare l'intera area-sistema della Carnia e della Val Degano. A questo proposito voglio qui richiamare una seconda considerazione. Oltre ai motivi storici già ricordati, va ribadito che le aspettative dei cittadini di Sappada sono assolutamente legittimate dal percorso che è stato seguito ai sensi del dettato costituzionale. Per questo territorio, infatti, valgono appieno i requisiti previsti dalla legge: la contiguità geografica, la stessa struttura economica e sociale, la vicinanza storico-culturale, così come è stato ricordato proprio dalla meritoria iniziativa della collega Isabella De Monte. E, cosa ancora più decisiva, vi è stata un'affermazione della volontà popolare univoca e chiara, al di là di ogni ragionevole dubbio. Tornerò tra poco su alcune criticità che legittimamente anche alcuni colleghi hanno espresso nel dibattito, ma credo sia assolutamente necessario riconoscere che quando i cittadini si esprimono con tanta forza, unità e determinazione, attraverso uno strumento riconosciuto dalla nostra Costituzione, sia obbligo del legislatore offrire una risposta adeguata e corrispondente alle aspirazioni democraticamente espresse. Potremmo - lo abbiamo fatto anche in occasione della riforma costituzionale - disquisire a lungo se un *referendum* sia sempre e comunque la migliore e più fedele modalità di rilevazione della volontà popolare, ma è certo che quando i cittadini si sono espressi è impossibile non tenerne conto. A questo proposito voglio agganciarmi, in conclusione, alla riflessione del collega Sonego che sottolineava ieri il rischio, oggi drammaticamente attuale alla luce della vicenda catalana, di affermare un principio unicamente nazionale e identitario nella definizione dei confini (in questo caso, confini regionali ma anche statuali). Dico al collega che la sua preoccupazione in termini generali è certamente anche la nostra, ma questo è un caso diverso, come ha ben richiamato il sottosegretario Pizzetti e che l'assoluta e trasversale unità di intenti dei cittadini di Sappada, la fondatezza della loro aspirazione, il pronunciamento favorevole, poi solo in parte ritrattato per strumentali contingenze elettoralistiche, dei Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, rendono assolutamente chiaro che non vi sono gli elementi di un uso distorto e potenzialmente conflittuale di questa vicenda. Una cosa va detta a questo proposito, anche a futura memoria. Credo che una diversa riflessione avrebbe con ogni probabilità fatto l'Assemblea del Senato se questa scelta avesse creato o fosse nata da strappi istituzionali, conflitti territoriali e rivendicazioni unilaterali non condivisi da maggioranze che, invece, potremmo definire quasi plebiscitarie, e se il riconoscimento della volontà dei sappadini non fosse stato così generale e trasversale. Poi, per fortuna, c'è l'Europa: le vicende di queste ore ci ricordano una cosa che dovremmo sempre tenere a mente e che vorremmo fosse di buon auspicio (è un augurio che esprimiamo per la soluzione positiva della crisi istituzionale che sta investendo la Spagna). Se è vero, infatti, che la condizione delle minoranze e delle specificità territoriali, la loro autonomia, il riconoscimento delle loro specificità e dei loro diritti, la loro tutela sono, come talvolta saggiamente diciamo, il miglior termometro del buon funzionamento di un sistema democratico, è altrettanto vero che la storia insegna che spesso, proprio in nome di malintese aspirazioni separatiste, strumentalizzando vicende tragiche di minoranze linguistiche e culturali, aizzando l'uno contro l'altro gruppi nazionali, obbligati in confini innaturali, il Novecento ha visto compiersi le peggiori nefandezze e i peggiori errori. Per questo crediamo che l'Europa, che altro non è - e dovremmo sempre ricordarlo - se non un insieme di minoranze, sia la cornice migliore entro la quale le giuste rivendicazioni a tutela dei gruppi minoritari e le diverse aspirazioni dei territori dovranno trovare sempre maggiore ascolto e anche, se possibile, una normazione generale, oggi affidata agli Stati nazionali. Proprio il comune contesto europeo è la migliore garanzia che tutto ciò diventi occasione di maggiore coesione e non motivo di divisioni e conflitti, che vogliamo lasciare definitivamente alla storia del secolo scorso. Per questo il Partito Democratico voterà a favore della proposta al nostro esame.

la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, che oggi voteremo, è un tassello ulteriore, dopo altri provvedimenti come quelli in materia di cinema e di spettacolo dal vivo, che segnano la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e una speciale attenzione alla formazione dei giovani. La grandiosità dell'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone è riconosciuta in tutto il mondo, a distanza di duemila anni dalla sua morte, come patrimonio comune. Il presente disegno di legge sottoposto all'esame della Assemblea è il frutto della sintesi di due disegni di legge e più precisamente dell'Atto Senato 2304, a prima firma della senatrice Pelino, e dell'Atto Senato 2355, a prima firma della senatrice Pezzopane. La 7a Commissione, addivenendo a un testo unificato, proposto dai relatori attraverso varie fasi in cui sono stati accolti sia emendamenti dei relatori sia emendamenti di varie componenti della Commissione, ha prodotto infine un testo finale largamente condiviso, che ha visto l'adesione ampia e trasversale delle forze politiche, grazie a tutta emarginata dai banchi dei licei perché estranea alla classica compostezza oraziana e virgiliana, caratterizzata da una vena passionale e anticonformista in contrasto con i valori tradizionali della Roma augustea, vena che fluisce libera e determina la modernità del poeta e dell'opera, si apre a una maggiore e più capillare conoscenza degli studenti, attraverso progetti e iniziative di enti pubblici e privati, in un programma di manifestazioni culturali nazionali e internazionali che promuovono anche la valorizzazione dei luoghi ovidiani. Sulmona, l'antica *Sulmo*, è la terra che duemila anni fa diede i natali al poeta elegiaco, il 20 marzo del 43 a.C.. Figlio di una famiglia facoltosa della classe equestre, a dodici anni si trasferì a Roma, insieme al fratello, per completare gli studi di grammatica e retorica. Ma non divenne retore: si sentì da subito incline alla poesia. Dopo una visita ad Atene, nelle città dell'Asia minore e in Egitto e il soggiorno di un anno in Sicilia, contrariamente alla volontà di suo padre si dedicò agli studi letterari, entrò nel circolo di Mecenate ed ebbe contatti stimolanti con i più importanti poeti del tempo: Orazio, Properzio, Virgilio. Produsse allora opere come gli Amores, le Heroides, i Remedia amoris, le Metamorfosi, i Fasti, ma soprattutto quello che fu il poemetto in distici elegiaci, opera della maturità che gli costò forse l'esilio: l'Ars amatoria. Siamo nel periodo storico della *pax augustea*, in cui i costumi e la morale, con l'influenza ellenistica, tendono a rilassarsi. Ovidio, il più giovane dei poeti elegiaci, rifiuta le contraddizioni del tempo, rifiuta i valori fissi e rigidi della vecchia società romana,

Nell'8 d.C. cade in disgrazia di Augusto ed è relegato nella lontana Tomi, oggi Costanza, nella Scizia, centro sul Mar Nero nell'attuale Romania.

Da qui continua a scrivere altre opere memorabili, come le Epistulae ex Ponto e, appunto, i Tristia. Nonostante il grande fervore letterario, l'autore non riuscirà mai ad ottenere, sino alla fine della l'agognato ritorno in patria. Si rivelarono del tutto inutili i suoi tentativi di convincere l'imperatore, prima Augusto, poi Tiberio. Morirà a Tomi il 17 d.C., senza avere mai più avuto la possibilità di rientrare nella terra natia. È quindi importante oggi,

Con questo atto s'intende rendere giustizia a Ovidio, onorarne la memoria, ma soprattutto valorizzare, tutelare e rimettere al centro dell'attenzione del mondo culturale e in particolare dei giovani la sua prestigiosa figura,

grazie a tutta finanziando negli anni 2017 e 2018 progetti di promozione, ricerca, salvaguardia e conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. In particolare, sostegno ad attività didattico-formative e culturali finalizzate a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; opera; il recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano; l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il museo ovidiano; grazie a tutta quale itinerario turistico-culturale; *e)* realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

ricerca. L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal presidente della Destinazione turistica di Sulmona-DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, Comitato promotore rimane in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione conclusiva nonché il rendiconto, quindi tutto all'insegna della massima trasparenza. È prevista l'istituzione di un comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità, che formulerà gli indirizzi generali per le iniziative di cui ai precedenti articoli.

In conclusione, ai componenti dei comitati non sono riconosciuti compensi (questo mi sembra importante), mentre i costi di funzionamento sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato

di Ovidio. L'articolo 4 prevede infine un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del Comitato promotore, per la predisposizione grazie a tutta

onorevoli colleghi, Publio Ovidio Nasone è il più moderno tra gli antichi, così potremmo definirlo. A lui si deve un'opera che, nonostante siano passati più di duemila anni, mostra ancora tutta la propria straordinaria attualità. Il provvedimento proposto all'Assemblea dalla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, che risulta dall'unificazione di due disegni di legge presentati, il primo all'inizio del 2016 dalla sottoscritta, si propone,

Il disegno di legge intende assicurare alla città di Sulmona, alla Provincia dell'Aquila e al territorio dell'intera Regione Abruzzo la possibilità di ricordare adeguatamente la figura e l'opera del sommo poeta. Si tratta di una ricorrenza di notevole rilevanza e di ampio respiro culturale, che certamente richiedeva un apposito intervento legislativo in grado di delineare la cornice delle manifestazioni, gli organi dedicati alla promozione promozione e alla formulazione degli indirizzi, nonché le risorse necessarie a realizzare una serie di importanti progetti. Sulmona, la provincia aquilana e l'Abruzzo saranno perciò al centro di una serie di iniziative culturali per la promozione dell'opera ovidiana e per il suo sviluppo. Sono varie e diverse le celebrazioni, soprattutto nella sua città, già iniziate e che stanno proseguendo durante questo 2017. Ci troviamo, infatti, in un centro dove si respira quotidianamente la presenza di Ovidio, una città che porta nel suo simbolo cittadino l'acronimo SMPE: «*Sulmo mihi patria est*», un verso tratto dai Tristia, una delle opere più decantate del poeta. A Sulmona, città che gli ha dato i natali, anche la biblioteca comunale e il liceo classico portano il nome del grande poeta. Ovidio è autore, tra l'altro, grazie a tutta grazie a tutta trasferitosi giovanissimo a Roma, dove studiò la grammatica e la retorica, ancor prima di dedicarsi alla poesia. Era stato esiliato nella odierna Costanza, in Romania, dopo essere caduto in disgrazia, sotto Augusto, a causa sembra di un *carmen*, che aveva colpito la sensibilità del primo imperatore romano Ars amatoria è il capolavoro della poesia erotica latina, dove il poeta elegiaco tratta dell'arte di amare, intrigando le donne romane dell'epoca, facendo innamorare molte matrone, tra cui, forse, anche Livia. E quell'interesse per lui da parte della terza consorte di Ottaviano Augusto fu forse la causa del suo esilio. Il disegno di legge prevede una serie di interventi da portare avanti durante quest'anno e durante il prossimo, 2018, al fine di promuovere la ricerca e la conoscenza della vita e dell'opera, ma anche dei luoghi in cui è vissuto Ovidio. Nei primi due articoli vengono delineate le finalità di sviluppo e promozione del patrimonio culturale culturale Ovidiano e il ventaglio di iniziative orientate al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, dando rilevanza all'opera e ai luoghi della figura ovidiana. Queste iniziative riguarderanno l'anno in corso e proseguiranno, appunto, nel 2018. Convegni, rievocazioni storiche, valorizzazione dei luoghi, manifestazioni di respiro culturale per diffondere ad ampio raggio l'opera del sommo poeta caratterizzano una stagione che porterà la città di Sulmona al centro dell'attenzione, nazionale e internazionale. E la promozione dovrà partire dai tanti progetti che sono già in corso e che si stanno sviluppando durante quest'anno. In tal senso dovranno essere promossi il recupero, il riordino e il restauro dell'opera artistica e del materiale storico, proprio allo scopo di ospitarlo in un museo di Ovidio, a tal fine individuato nella città di Sulmona. Anche la riorganizzazione e, ove necessario, il recupero edilizio, dei luoghi in cui Ovidio ha vissuto e ha scritto, sia a Sulmona che nella Valle Peligna, rientrano nelle finalità di questo disegno di legge, che si propone inoltre di istituire un parco letterario ovidiano, costituendo un nuovo itinerario turistico e culturale. Viene altresì prospettata una serie di gemellaggi tra le città che ospitarono Ovidio:

in materia di studi ovidiani. Le ricerche vengono inoltre promosse per favorire l'eventuale individuazione e pubblicazione di materiali inediti del grande poeta. Per coordinare quello che si auspica un vasto lavoro di celebrazioni ovidiane, viene istituito, dalla presente legge, un comitato promotore, composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dei beni e delle attività oltreché dal Presidente della Regione Abruzzo e dal sindaco di Sulmona al fine di valorizzare la figura di Ovidio. Un comitato scientifico, istituito dal comitato promotore e composto da massimo dieci personalità della cultura e dell'arte letteraria latina, avrà il compito di formulare gli indirizzi generali delle iniziative indicate. Vi sarà anche un comitato di giovani studiosi di venticinque anni) che avrà il compito di formulare proposte al comitato promotore. Questi giovani studiosi saranno selezionati con apposito bando del Ministero dell'istruzione. Ovviamente, lo scopo di questo provvedimento è anche quello di favorire una maggiore diffusione internazionale dell'opera e del pensiero del poeta latino. Al disegno di legge è affidata una dotazione non eccessiva, ma simbolicamente adeguata, di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla dotazione riservata degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Noi ci impegniamo ad essere di sprone e di controllo, affinché quella dote finanziaria venga utilizzata al meglio e ponga le basi per proseguire questo anno ovidiano anche nei prossimi anni, come invito a progredire nello studio e nella celebrazione della modernità di un grande poeta antico, indissolubilmente legato alla sua città natale, Sulmona.

Il primo aspetto è l'importanza in termini culturali dell'opera di Ovidio. Egli è profondo conoscitore della lingua latina e della lingua greca e per questo leggere Ovidio oggi significa attingere direttamente da una delle fonti più ricche della cultura antica e, quindi, della cultura occidentale. Scrittore fondamentale dell'epoca augustea insieme a Virgilio e Orazio, Ovidio è poeta a tutto tondo sia perché fin dalla sua formazione decide di abbandonare il *cursus honorum* politico per dedicarsi a tempo pieno all'attività di scrittore sia perché, nel corso della sua prolifica attività letteraria, sperimenta quasi tutti i generi poetici, raggiungendo sempre

Ed è proprio sulle Metamorfosi che vorrei porre l'attenzione nella analisi del secondo aspetto legato all'importanza di Ovidio, come poeta della memoria culturale. Le Metaforfosi, infatti, non sono semplicemente un'opera antologica in senso stretto, ma prima di tutto una rielaborazione del sapere greco in chiave latina. Ovidio è un consapevole rielaboratore del passato: fa tesoro della cultura greca ellenistica, che a sua volta si era fermata a ragionare sulla cultura greca classica, e tesse le lodi del passato usando come chiave di racconto la mitologia. La consapevolezza è tanto più chiara se si pensa all'opera come ad un erudito e programmatico dialogo con il passato da parte di un presente che stava vivendo in quel momento un mito moderno. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma, dopo tanti anni di lotte fratricide che avevano ridisegnato le egemonie nel Mediterraneo, proprio negli anni di massima attività del poeta, realizza il sogno di una pace universale che unisce tutta la cultura allora conosciuta sotto l'egida romana. Troviamo dunque nelle Metamorfosi la *summa* enciclopedica della cultura greco-latina e la testimonianza storica di un'epoca d'oro. Ma non è tutto. Il terzo aspetto per il quale Ovidio è una figura di riferimento necessaria per la nostra cultura è che egli è poeta del futuro e con Le metamorfosi disegna un progetto culturale che è destinato ad attraversare i secoli. Egli, infatti, prima di tutto individua un tema che è alla base di ogni suo racconto: il cambiamento. Il cambiamento è per Ovidio, e grazie a lui anche per noi, una nuova filosofia del sapere. La metamorfosi è intesa come approccio metodologico alla ricerca: la consapevolezza che tutto è destinato a cambiare, nella sua forma, ma non nella sua sostanza. Questo è il cuore pulsante dell'opera ovidiana, ed è questo che oggi lo rende uno degli scrittori antichi più attuali. Il suo insegnamento è tanto più forte quanto più si allontana dalle contingenze storiche per raggiungere la ricerca della natura umana. I personaggi ovidiani infatti, anche se spesso sono semidei, fauni e ninfe, sono in definitiva forgiati con una profondissima umanità. I loro cambiamenti sono spesso dolorosi e irreversibili, ma mai inconsapevoli: questo è il concetto che voglio approfondire. Sono sempre il frutto di una scelta che Ovidio pone come prerogativa imprescindibile nei suoi racconti: sapere da dove veniamo ci dà la libertà di scegliere dove vogliamo andare, senza per forza scegliere il meglio per noi. Questo è un concetto importantissimo. Ad Ovidio è sufficiente, infatti, una scelta consapevole ed è la consapevolezza a permetterci la libertà.

grazie a tutta La civiltà romana, seppur in un'ottica imperialista, ebbe fin dalle sue prime conquiste territoriali l'intelligenza di rispettare e fare tesoro delle culture dei popoli che conquistava, primo fra tutti il popolo greco. L'unione politica romana è stata resa possibile per oltre mille anni a partire dal rispetto delle culture del Mediterraneo: un dialogo, questo, che ha portato allo sviluppo della moderna cultura occidentale. Il provvedimento che oggi stiamo discutendo, con le misure rivolte ai giovani studiosi e al settore dell'istruzione (sono già state elencate), si iscrive a pieno titolo nella direzione auspicata da un ordine del giorno che abbiamo approvato in 7a Commissione (approvato anche dal Governo), durante la discussione dell'Atto Senato 2371, Nel dispositivo leggiamo al primo punto leggiamo al primo punto un impegno al Governo «a farsi garante di una continua sensibilizzazione soprattutto nelle politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta delle lingue latina e greca, come massima espressione della sostanza culturale d'Europa, portata in diverse parti del mondo». L'Europa tutta, infatti, riconosce nelle civiltà greca latina le radici storiche del proprio mondo e il tesoro inesauribile della memoria comune del vecchio continente. Un'importante risposta viene data proprio da questo disegno di legge e il Governo

conseguente alla legge n. 107 del 2015, alla citata legge n. 44 del 2017, ma anche la Convenzione di Farola, la cui ratifica ci aspettiamo sia portata al più presto in questa sede, che porta all'attenzione soprattutto il discorso della memoria e dell'eredità. Auspichiamo inoltre che il presente disegno di legge sia al più presto approvato in via definitiva per dare ragione dell'operatività progettuale che è già in atto e che è stata ricordata dalle colleghe e consentire un'operazione che

che specificamente il territorio da cui proviene la proposta ha dovuto fronteggiare in questi anni. La valorizzazione di questi luoghi, simbolo della vita di Ovidio, come la città di Sulmona che gli ha dato i natali, sono proprio il rafforzamento dell'identità culturale

infatti che ci sono ancora materiali inediti. Abbiamo parlato dunque di Ovidio come conoscitore della lingua e della cultura grecoromana, come poeta della memoria culturale e filosofo del cambiamento. Concludo osservando come alla base di questi aspetti si debba considerare Ovidio figlio di una cultura matrice di tutte le culture, che non va annichilita nella considerazione di una cultura passata, ma alimentata con lo stesso nutrimento con cui Ovidio nutriva i suoi personaggi: l'attenzione per l'uomo.

anni dalla morte di Gioachino Rossini e così tutte le altre. Le risorse stanziate per il funzionamento dei relativi comitati promotori e per il finanziamento dei progetti valutati sono derivati dai capitoli di spesa nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già alimentati in forma stabile con apposita norma inserita in legge di bilancio.

che può essere ben annoverato in termini comparativi, almeno rispetto al resto dei Paesi europei, come quello con la maggiore densità territoriale di beni culturali. Nel caso dei disegni di legge in esame stiamo parlando di un impegno di spesa di 700.000 euro complessivi per le celebrazioni di Ovidio, 700.000 euro complessivi per le celebrazioni di Gioachino Rossini e 3.450.000 euro grazie a tutta in esame sarà dunque certamente favorevole, perché la cultura, soprattutto quando fortemente alimentata da iniziative tese a salvaguardare la memoria la figura di illustri personaggi, con particolare attenzione ai programmi che saranno svolti, è sempre un fattore positivo di crescita per i nostri ragazzi, uomini e donne di domani. Non posso però non stigmatizzare il fatto che per circa 240.000 studenti disabili delle scuole italiane tali iniziative non saranno pienamente accessibili per la carenza endemica di docenti di sostegno, problema, questo,

tengano nella debita considerazione quelli che si rivolgono, coinvolgono e favoriscono la partecipazione di studenti disabili. La cultura è infatti un diritto di tutti, nessuno escluso, e non può, né deve incontrare impedimenti, neppure la carenza di insegnanti di sostegno. Da ultimo, ma non per ultimo, vorrei fare un'osservazione.

Ci vorrebbe sì la cultura: introduciamo cultura del rispetto. Abbiamo l'emergenza della povertà, con la necessità, anche qui, di cultura, della cultura della condivisione. Abbiamo emergenza di democrazia

non solo a quella del ricordo e della storia delle sue arti, ma anche a quella dell'accoglienza e dell'inclusione. Se vogliamo che i nostri figli accettino i disabili a scuola, dobbiamo educarli a considerare sempre gli ultimi e a pensare

è una giornata un po' particolare, perché approviamo un provvedimento che sostiene le celebrazioni ovidiane ed è un giovedì mattina qui, nel Senato della Repubblica, parliamo di cultura, ricordando una figura eminente della nostra storia e letteratura. Siccome c'è anche una scuola superiore, ho inteso prendere la parola perché, tra i vari aspetti importanti che sono stati sottolineati del pensiero di Ovidio (il più moderno degli antichi, come ha detto la senatrice Pelino, e il poeta della memoria, come ci ha ricordato la senatrice Elena Ferrara) ci sono due parole sulle quali vorrei riflettere insieme a voi. Sono parole che sono state graffite su un muro di Ercolano,

probabilmente era un messaggio trasversale di tipo elettorale, ma anche una velata minaccia, rivolta a un cittadino di Ercolano, che, candidandosi a una carica pubblica, doveva mettere in conto di essere ossequiente al potere, altrimenti rischiava di fare la fine di Ovidio, «morirai a Tomi». È importante ricordare in quest'Aula, nel Parlamento italiano, che chi ambisce a rappresentare la cosa pubblica deve, da un lato, rifuggire ogni tentativo di pressione indebita sulla sua attività e, dall'altro, avere come esempio figure eccezionali come Ovidio, che fu non solo un grande poeta, ma anche una persona inserita nella vita del suo tempo: apparteneva all'ordine equestre, ma non ambì mai al laticlavio, volendo mantenersi libero e non succube di un potere che, al suo tempo, era particolarmente permeante e invasivo, quello di Augusto. Partecipava piuttosto al circolo di Messalla Corvino e non a quello di Mecenate e forse questa sua indipendenza intellettuale - lo dico ai ragazzi che sono presenti in tribuna - gli costò l'esilio a Tomi, Tomi, dal quale non ritornò mai e che lo rende, tra i grandi della letteratura latina, uno dei più grandi per la dirittura morale e la capacità d'interloquire con il potere, restando sempre coerente con i suoi principi ideali. Mi fa piacere che nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, se l'Assemblea lo riterrà, siano incluse anche borse di studio per incoraggiare i nostri giovani ad approfondire il pensiero di Ovidio, grande letterato, ma davvero grande cittadino romano e dunque esempio illustre da ricordare in quest'Aula

Signora Presidente, evidentemente pochi hanno raccolto l'invito fatto in precedenza. Mi offro volontaria per passare

impegna il Governo ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale

allora siccome l'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di spingere il Governo a cercare risorse aggiuntive, sono sono disposta ad "epurare" il testo di tutte le parti politicamente rilevanti, perché è questo quello che mi si sta chiedendo di fare, nel senso che mi si sta chiedendo di togliere le riflessioni politiche all'interno di questo ordine del giorno, al di là della correzione tecnica.

grazie a tutta ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura del poeta abruzzese. Tale compito spetta al legislatore statale, perché le specifiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell'ambito delle finalità di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazionale, come quella contenuta nella proposta che ci accingiamo a votare, devono essere garantite esclusivamente dalla legge statale. Più in generale, la proposta contenuta nel testo riguarda un bene comune per eccellenza, la conoscenza. Essa rappresenta un beneficio per tutti, un gioco a somma positiva, poiché di essa ci si può nutrire assieme senza che il consumo di un singolo escluda dal godimento un altro consociato. Il nostro impegno deve tendere a garantire non solo l'informazione, la corretta ed esaustiva rappresentazione dei fatti, della vita e delle opere di Ovidio, bensì anche un obiettivo ancor più perché più elevato: fornire a chiunque, in particolare agli studenti, la possibilità di possedere un insieme di informazioni organiche, organizzate ed elaborate per poter apprendere e diffondere la comprensione e l'esperienza derivanti dalla conoscenza della cultura ovidiana. Accogliamo con piacere quindi il provvedimento, con un plauso particolare per la parte in cui esso mira a garantire il sostegno ad attività didattico-formative e culturali per promuovere, in Italia e all'estero, la consapevolezza dell'importanza della vita e dell'opera di Ovidio. Analogamente virtuosa appare la strada intrapresa per raggiungere l'obiettivo, ovvero la strada della «collaborazione con enti pubblici e privati» per la realizzazione delle «attività didattico-formative e culturali». Il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato è auspicabile, non solo perché rispondente al contenimento della spesa per investimenti, all'ottimizzazione dei costi operativi, al riconoscimento

sotto il profilo delle soluzioni organizzative in grado di favorire una corretta amministrazione e promozione del settore stesso. Concludiamo con l'apprezzamento di un'ulteriore previsione contenuta nella norma. Ci riferiamo al fatto che il comitato promotore sia composto non solo da cariche apicali dell'Esecutivo stesso, oltre che da «personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio», ma anche da un comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani». L'obiettivo ambizioso, che mira a raggiungere obiettivi importanti e concreti, come la promozione della conoscenza, in Italia e all'estero, della vita e dell'opera di Ovidio, il recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, il recupero edilizio e la riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, la costituzione di un parco letterario ovidiano e la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti, è da noi condiviso. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà al provvedimento in esame. Signora Presidente, colleghi, discutere questo disegno di legge ci offre la possibilità di approvare sì un'ottima iniziativa delle senatrici Pelino e Pezzopane, che con Ovidio condividono di certo i natali, ma al contempo ci offre la possibilità di celebrarlo a anni dalla scomparsa e di prendere spunto dalla sua straordinaria vita e dalle sue illuminanti opere per cogliere l'occasione di soffermarci su diverse riflessioni. L'iniziativa legislativa in merito a una commemorazione così importante si è resa necessaria per fare in modo che tutti possano riscontrare come la genialità del poeta nelle nostre classi scolastiche, quelle che

dalla classica compostezza dei suoi tempi. Forse le insegnanti o gli insegnanti lo conoscono poco, quindi è difficile portare nelle scuole un autore poco o mal conosciuto. conosciuto. A duemila anni di distanza trascuriamo colui che fu, oltre che un poeta di grandezza smisurata, un rivoluzionario, un anticonformista, un precursore. A duemila anni di distanza tendiamo a non evidenziare le gesta, oltre che la poesia, di uno dei più grandi italiani; un uomo che duemila anni fa scrisse le Metamorfosi, testo abnorme e stupefacente creazione letteraria; un poema epico nel quale Ovidio ha raccolto tutto lo scibile umano e nel quale però non ha taciuto le verità di una realtà sociale che lui stesso ha vissuto fuori dalle righe. righe. A duemila anni di distanza questo sembra ancora disturbarci e, come purtroppo spesso è accaduto, lo ha portato all'esilio. le Metamorfosi (a mio parere già il titolo non poteva essere più rivoluzionario) Ovidio racchiude tutte le brutture e le bellezze dei percorsi della vita. In essa Ovidio sviscera e non nasconde gli aspetti della vita come come l'amore in quanto tale e in tutte le sue forme (la gelosia, l'invidia, la cattiveria, la mancanza di meritocrazia, la tirannia)

Belpaese si sconvolgerebbe: ciò è lezione del fatto che non sono gli anni ma le menti che portano all'evoluzione sociale.

lo portarono in esilio, quindi lo allontanarono negandogli la possibilità di arricchire con il suo pensiero e le sue ragioni il popolo tutto. Lo abbiamo fatto con Dante, che è considerato solo il padre della lingua italiana: anch'egli, contrastato per la sua vita strettamente legata agli avvenimenti della politica, politica, fu esiliato e non rivide mai più la sua patria. Tra l'altro ho l'onore di vivere nella terra della Lunigiana che lo ha ospitato in esilio per due lunghi anni e dove ha scritto i meravigliosi canti del Purgatorio, descrivendo il paesaggio di quella splendida terra. Lo abbiamo fatto con Machiavelli che, spinto dalla possibilità di salvarsi e compiacere chi lo poteva graziare dal suo esilio, scrisse proprio in esilio la sua opera maggiore, Il Principe. Ebbene, lo abbiamo fatto per Bettino Craxi, ultimo statista italiano dal quale il Paese ha preso il meglio, con cui l'Italia ha raggiunto la vetta dei Paesi più industrializzati, la dimensione che la politica dovesse essere anticonformista; eppure il Belpaese, dopo aver preso il meglio che egli potesse dare, lo ha lasciato morire in esilio. Tutti sanno che quello è stato uno dei pochi tentativi di cambiare davvero il sistema politico e il nostro Paese, ma pochissimi lo dicono, anche a distanza di anni, e quindi tentano di manipolare la storia.

Credo che oggi stiamo investendo più che bene il nostro lavoro in Assemblea per far sì che la commemorazione di Publio Ovidio Nasone diventi legge, poiché credo fermamente che questo la nostra Italia, debba necessariamente investire e fare in modo che gli strumenti culturali diventino parte pregnante della nostra società. Ovviamente devo ripetere al Governo che è necessario "svecchiare" i nostri docenti, insegnanti giovani nella scuola. La visione delle cose e delle diversità non deve mai essere adombrata da sterili preconcetti, ma deve essere illuminata, sebbene non condivisa, affinché il Paese impari ad avere un'analisi oggettiva oltre che di massa. I populismi non servono a nulla se non a portare i nostri uomini migliori in esilio. In questo, tutti devono fare la loro parte: la politica, che deve pensare sempre e comunque al bene del Paese, senza lanciare ai cittadini false esche, portandoli a conoscere conoscere molti *slogan* e pochi fatti; l'informazione, che ad esempio non può continuare ad avere la presunzione di condurre i processi sui giornali, demolendo le vite di persone che la nostra Costituzione vuole innocenti fino al terzo grado di giudizio, esiliandole a non poter continuare la loro vita poiché marchiati da un'opinione pubblica che si sta allenando a non fare sconti a non avere indulgenza, anzi. Ma la parte più importante la devono fare i nostri insegnanti, la nostra scuola, i nostri programmi scolastici, sia pubblici che privati,

tutti i mezzi per poter scegliere chi essere.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, a nome di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, esprimo il nostro consenso al disegno di legge che istituisce l'anno ovidiano e le celebrazioni della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, com'è stato ricordato, l'immortale autore delle Metamorfosi, straordinaria raccolta di miti di trasformazione: uomini che diventano animali, piante, statue, girasoli, ragni, pipistrelli, forse anche (non ricordo) uomini di destra che diventano di sinistra e uomini di sinistra che diventano di destra. Farlo proprio oggi mi sembra particolarmente significativo. È infatti questo il giorno in cui al Senato viene presentata in Commissione una nuova legge elettorale, il Rosatellum o il Trasformellum che dir si voglia, che, nel caso in cui fosse approvata, istituzionalizzerebbe il trasformismo completando la metamorfosi italiana. Nel nome del venerando Ovidio che celebriamo ci opporremo, come si diceva una volta, ma lo faremo nel Parlamento e nel Paese. Oggi sosteniamo questo disegno di legge a lui dedicato, che prevede di far conoscere agli studenti l'opera di Ovidio e un programma di manifestazioni culturali nazionali e internazionali che promuovono la giusta valorizzazione dei luoghi ovidiani, ma con lo spirito che ho voluto condividere con l'Assemblea.

Ricordo che siamo partiti da due disegni di legge, di origini abruzzesi, per così dire, in seguito unificati per perseguire un obiettivo comune: diffondere la conoscenza e approfondire lo studio delle opere di Ovidio. Con questo provvedimento si immagina di intraprendere una serie di azioni e iniziative, sia pubbliche che private, nel quadro di un programma di manifestazioni culturali, nazionali e internazionali, che promuovano anche la valorizzazione dei luoghi ovidiani. Tali progetti appaiono quanto mai opportuni, poiché l'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone ha segnato profondamente la cultura e la storia dall'epoca romana fino ai nostri giorni. Sicuramente riconosciuto come uno dei più grandi poeti latini, Ovidio è ancora studiato nelle più prestigiose università del mondo per modernità e attualità di linguaggio e contenuti. Questo proprio per una lirica caratterizzata da passionalità sincera e senza costringimenti stilistici, che ne hanno subito fatto un poeta rivoluzionario ed innovatore. Il provvedimento mira a sfruttare la ricorrenza dei duemila anni dalla morte del grande poeta per celebrarne la figura e le opere, contribuendo alla massima diffusione internazionale dell'opera e delle conoscenze legate ad esso. All'articolo 2 si elencano gli interventi da intraprendere. I progetti previsti sono da attuare sia nel 2017, anno ovidiano, sia nel 2018 e comprendono il sostegno ad attività didattico-formative e culturali; il recupero e il restauro del materiale storico e artistico ovidiano e dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, a Sulmona o nella Valle Peligna; la costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale e di un museo dedicato ad Ovidio, nella città di nascita; infine, un gemellaggio istituzionale tra quest'ultima e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. Si prevede opportunamente che tali attività dovranno essere coordinate da un comitato promotore, in carica fino alla fine del 2018, che comprende rappresentanti del Governo, della Regione Abruzzo e della città di Sulmona, oltre a personalità esperte della materia. L'azione del comitato promotore sarà ispirata e monitorata da un apposito comitato scientifico. A questi due organi si aggiunge, con funzione consultiva, un comitato di giovani *under* venticinque, studiosi dell'opera ovidiana, denominato «Comitato dei cinquanta «Comitato dei cinquanta ovidiani». Tutte le attività del disegno di legge sono finanziate con un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ovidio rappresenta ancora oggi uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, con la sua vitalità intellettuale inesauribile. Il Medioevo lo considerò non inferiore a Virgilio ed ebbe inoltre notevole influenza su tutta la poesia umanistica italiana e sullo stile dotto e sui carmi dei filologi franco-olandesi. È quindi importante che l'Italia ricordi questo grande scrittore e compositore poetico che ha dato lustro alla Penisola in tutto il mondo. La storia di un popolo passa anche dalla protezione e valorizzazione della propria cultura che, con il presente provvedimento, si cerca di tutelare, consegnando ai posteri la prestigiosa Siamo sicuri che i progetti presenteranno ampi e qualificati livelli di collaborazione fra istituzioni, scuole e privati, sul piano nazionale e internazionale, valorizzando anche singole e autonome proposte a livello locale o di singole città. Si creerà un sistema virtuoso, che congiungerà l'ottimizzazione delle risorse, la qualità delle proposte, il coordinamento dei calendari e delle attività di promozione sul piano nazionale e internazionale. Gli obiettivi di promozione, ricerca, salvaguardia e conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio potranno essere raggiunti con interventi di messa a punto e potenziamento delle strutture e delle istituzioni già esistenti e attive sui luoghi ovidiani. In conclusione, un Paese che ricorda il proprio passato può aspirare a diventare o confermarsi guida di tutela e celebrazione storico-letteraria a livello internazionale. Un Paese che valorizza adeguatamente l'opera dei propri cantori più autorevoli, fondatori di quella cultura classica alla base della nostra anima italiana, può trovare la giusta strada per formare le nuove generazioni e, quindi, il proprio futuro. Il provvedimento al nostro esame contiene gli strumenti per procedere in quelle direzioni. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa popolare-Centristi per l'Europa.

in difficoltà. Da un canto, riconosciamo l'altissima valenza che un provvedimento del genere rappresenta: la promozione della cultura e di quella ovidiana in particolare, in un territorio che ha bisogno di ripartire, di crescere e anche di rinascere. E quali, se non i canali culturali,

che sicuramente vanno migliorati. Il tema dei finanziamenti è stato già affrontato in sede di esame degli emendamenti. Abbiamo visto che il Governo si è impegnato

degli archivi e delle biblioteche statali; ci fu anche un appello firmato da tante persone, tra cui studiosi ed intellettuali - ricordo Eco, Montanari, Magris per cercare di salvare questi istituti. A quanto pare ci siamo riusciti nel corso della legislatura, ma purtroppo, una volta salvati, si comincia di nuovo ad usarli come serbatoio

Ancora una volta, in questo comitato si fa anche la confusione tra organi consultivi ed organi esecutivi: c'è un comitato scientifico, ma alcuni suoi membri sono anche componenti del comitato promotore. In realtà sarebbe più sano separare nettamente la fase consultiva e propositiva dalla fase esecutiva, in modo tale che ci possa essere un bilanciamento e un monitoraggio, ancora più efficace, tra questi due organi, che dovrebbero essere indipendenti

Anche il tema del monitoraggio e del controllo rimane aperto. Il comitato promotore pubblica sul proprio sito istituzionale la relazione conclusiva, ma un vero

ha un problema di ripartenza, un problema di sottosviluppo in alcune Regioni e, in particolare, nel Meridione. Perché allora non affrontare questo tema, che è strategico da un punto di vista più generale? Occorrerebbe predisporre un piano di intervento culturale,

grazie a tutta grazie a tutta

grazie a tutta

esserlo avrebbe significato non riconoscere la sua originale e straordinaria vena poetica. L'estrema facilità di composizione di cui Ovidio era dotato non sconfinò mai nel banale verseggiare, ma fu invece il suo punto di forza, il suo carattere distintivo, l'autentica e l'alta dimostrazione di quella immediata espressione del sentimento che è la poesia. La sua opera va ben oltre le Metamorfosi citate oggi in Assemblea. Se l'intenzione è valorizzare, far conoscere a tutti e trasmettere ai giovani il nostro patrimonio e la nostra identità culturale, ben vengano iniziative come questa in Assemblea, in cui si discute di cultura, letteratura e opere letterarie, che sono la storia del nostro Paese. Sarebbe auspicabile un intervento normativo più organico, come è stato richiesto nell'ordine del giorno approvato, a prima firma della collega Montevecchi. Ovidio è nato a Sulmona e per noi abruzzesi è un orgoglio, un punto di riferimento irrinunciabile.

internazionale. Vi sono, quindi, non solo l'intenzione di celebrare una ricorrenza, quella appunto dei duemila anni dalla sua morte,

un approccio lodevole che si rinviene in modo inequivocabile nella ferma intenzione di sviluppare una seria attività di ricerca intorno all'opera del grande poeta abruzzese, finalizzata soprattutto alla raccolta di materiali ancora inediti. Il disegno di legge in esame prevede una copertura finanziaria di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e definisce gli obiettivi che devono essere perseguiti totale condivisione dal comitato promotore e dal comitato scientifico: sviluppo di iniziative finalizzate al sostegno delle attività didattico-formative di promozione dell'opera ovidiana; il recupero, il restauro e il riordino del materiale storico e artistico dell'opera di Ovidio, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitarne il museo; il recupero dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona, sia nella Valle Peligna; la costituzione di un parco letterario ovidiano quale itinerario turistico-culturale; la realizzazione di un gemellaggio tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo di soggiorno e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, attraverso la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

Tali obiettivi sono sicuramente condivisibili e mi auguro che il loro raggiungimento abbia ricadute economiche, occupazionali e turistico-culturali importanti, per la Provincia aquilana e l'intera Regione Abruzzo. Non si comprende però la ragione per la quale nel comitato promotore, oltre alla condivisibile partecipazione del sindaco di Sulmona, si debba dare spazio al Presidente della Regione Abruzzo e a due parlamentari del territorio. In questo modo, cari colleghi, si corre concretamente il rischio di dimenticare i buoni propositi del disegno di legge che ho enunciato, facendoli passare in secondo piano, e di contribuire ad alimentare la sensazione, per altro ormai diffusa, che la politica cerchi in tutti i modi di mettere il cappello su ogni progetto. È per questo che molte persone possono provare fastidio e considerano inutili e strumentali questi provvedimenti, anche a fronte dei concreti e cogenti problemi che i cittadini vivono quotidianamente.

grazie a tutta

la figura e la grandiosità dell'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone. La sua intelligenza e la sua eccelsa genialità poetica hanno segnato profondamente la cultura e la storia, dall'epoca romana sino ai nostri giorni. È un'occasione straordinaria e irripetibile per ricordare all'Italia e a tutto il mondo le qualità poetiche di Ovidio, a distanza di duemila anni dalla sua morte, come patrimonio dell'umanità. Con l'auspicio che l'*iter* prosegua velocemente alla Camera e che diventi legge un testo con un finanziamento non eccessivo, ma utile a coadiuvare le tante iniziative già messe in piedi in sede locale dal Comune di Sulmona,

sull'anno ovidiano con forte autorevolezza, per far capire a tutti che non stiamo facendo un regalo o un obolo a una comunità, che così magari organizza qualche iniziativa festosa, ma stiamo dentro un tracciato che il Governo ha messo in campo e che rimette in moto processi di alto valore culturale.

si è tornati a reinvestire nella cultura e a un impegno finanziario che va oltre i due miliardi, con la legge sul cinema e gli altri provvedimenti che bene la presidente Di Giorgi ricordava durante il dibattito sul disegno

un ritorno, all'interno di un progetto complessivo che magari aiuta anche a promuovere il turismo sulla base dell'alta valenza culturale di un passato che parla al futuro.

In realtà Augusto, quando decise di mandar via da Roma il grande Ovidio violò alcune regole. La *relegatio*, infatti, in base al diritto romano, andava inflitta a seguito di un pubblico processo e doveva essere ratificata dal Senato, ma ciò non avvenne. L'imperatore dittatore decise da solo: Ovidio va via da Roma e non ci torna più. Oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge, pur simbolicamente, facciamo ritornare ufficialmente il poeta, cantore dell'amore, qui a Roma, qui in Italia, a tutto campo e a tutto titolo. I luoghi di Ovidio, nella terra di Ovidio, sono importanti. Ricordiamo che lì c'è il tempio di Ercole Curino, c'è la *fons* *amoris*, ci sono i resti della villa di Ovidio. C'è una splendida montagna, una Conca Peligna, con Sulmona al centro e i monti che fanno corona. C'è la Badia Morronese e, proprio proprio salendo su quella strada per le marane, si raggiunge Fonte d'amore, la fontana celebrata da Ovidio. All'ombra di quegli alberi risuonano i versi ovidiani, tratti da Tristia, che prima venivano ricordati: «*Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, milia qui novies distat

Il 2017, con questo disegno di legge, viene dichiarato anno ovidiano. Ho ricordato quei luoghi di Sulmona perché proprio in quei luoghi per settimane è divampato un incendio criminale e proprio in quei luoghi si sono sfidate le forze più positive. Ed è sempre a Sulmona che a dicembre si è dovuto ricordare con dolore, alla presenza delle alte cariche dello Stato, la morte della giovane Fabrizia Di Lorenzo, colpita da un atto terroristico a Berlino. Cito questo perché voglio far capire che con questo atto importante diamo a quella terra un segno di qualità e di valore, una sorta di sorta di opportunità. Le celebrazioni sono già iniziate, l'attesa per questa legge era tanta ed ora noi rispondiamo

Le celebrazioni sono iniziate e con questo disegno di legge potranno avere un forte sostegno. Sentivo alcuni colleghi preoccupati per i controlli, ma cosa c'è di più autorevole, nei controlli, della Corte dei conti e della procura della Repubblica? Perché, nell'atto di formulare una legge avanzata, che dà ai territori tante opportunità, dobbiamo già da subito criminalizzare quei territori? Se ci saranno problemi, se ne occuperanno le autorità competenti, ora noi facciamo il nostro lavoro, che non è certo quello di pensare pregiudizialmente che quelle risorse possano essere distolte, ma semmai di dare degli strumenti positivi perché quelle risorse, come abbiamo fatto,

per quei ragazzi abbiamo previsto una norma specifica. Ovidio diceva: «Lodiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri». È questo il messaggio che diamo a quei giovani: mentre lodiamo i tempi passati, vogliamo dar loro gli

la struttura perché, come sapete, la Regione Lombardia ha messo a disposizione il palazzo dove potrebbe trovare sede l'EMA in forma gratuita, almeno per il primo anno. anno. Allora, poiché c'è una grande volontà del Paese e anche un interesse che questa agenzia possa venire in Italia, vorrei sollecitare affinché la mia mozione sia messa in discussione al fine di poter dare un contributo anche parlamentare

una calendarizzazione celere proprio perché così il *Premier*, i Ministri e chi sarà deputato a difendere la candidatura, possano essere forti di una decisione parlamentare. Ricordo i tempi: a fine mese avremo la scrematura dalle 19 sedi proposte; poi, dal 20 ottobre al 20 novembre la votazione. A tal fine si è costituito anche un gruppo interparlamentare con

per sapere quanti fossero gli alunni disabili presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, di quante ore di sostegno necessitassero e quante di queste fossero coperte da insegnanti di sostegno. Tali dati venivano chiesti suddivisi per Provincia e Regione. La richiesta è stata presentata nel 2014 e nel 2015; la risposta è sempre stata parziale: sembrerebbe che non si possa rilevare centralmente l'orario effettivo di sostegno assegnato a ogni singolo studente, a detta del Sottosegretario. Esiste dunque un vuoto, certamente colmabile, nelle procedure di rilevazione dei dati di rilevazione dei dati da parte del Ministero. Secondo il MIUR quest'anno gli alunni disabili sono più di 234.000, molti dei quali (uno su tre) non avranno un insegnante di sostegno di ruolo, a discapito della continuità didattica prevista per legge, perdendo così ogni anno un punto di riferimento scolastico e affettivo. Gli studenti disabili hanno diritto all'istruzione come tutti. Una sentenza della Corte costituzionale (la n. 275 del 2016) recita: «È la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione». Continuerò in questa sede a ricordare questo baco fintantoché non avrò una risposta in grado di

da una base sovietica partì l'allarme che cinque missili con testate nucleari erano partiti dagli Stati Uniti e si stavano dirigendo in Russia per colpirla. Ora, se ci fosse stato un qualsiasi funzionario, qualsiasi militare, questa storia sarebbe finita nel peggiore dei modi con l'olocausto nucleare perché il militare avrebbe semplicemente avvisato il Cremlino - nel 1983 i rapporti tra USA e Russia erano pessimi - e il Cremlino avrebbe dato l'ordine per il lancio dei contro missili verso gli Stati Uniti

il Papa è una figura che sta facendo più di tutta la politica mondiale messa insieme. Ricordiamo, tra l'altro, che la Corte di giustizia dell'Aja

Grazie dal punto di vista dell'impegno nello smantellamento delle armi nucleari. Vorrei ricordare che, molto cinicamente, dal punto di vista economico, mantenere, manutenere e aggiornare i sistemi d'arma nucleare ha un costo talmente elevato, che se si utilizzassero queste risorse per combattere la fame nel mondo,

Signora Presidente, oggi è il 21 settembre, la Giornata mondiale dell'Alzheimer. Questa è un'occasione molto importante per riflettere su una realtà che sono in Italia colpisce oltre 600.000 malati, destinati ad aumentare, anche perché il nostro è il Paese più longevo d'Europa, con quasi 14 milioni di ultrasessantenni. Si tratta di una patologia per cui ancora non ci sono cure definitive e che riverbera, tra l'altro, i suoi cupi riflessi non solo sul malato, ma anche su chi gli è vicino, come pochissime altre malattie. Esso diffonde infatti sensazioni come depressione, impotenza e disperazione. L'Alzheimer è una malattia molto personalizzata: c'è chi resta in silenzio e c'è chi invece sproloquia verso i suoi interlocutori, molto spesso immaginari, usando di volta in volta infermieri, badanti o familiari come destinatari prescelti di questi loro sproloqui. Ognuno ha il suo delirio e per ognuno c'è una sorta di ritorno all'infanzia. Il morbo di Alzheimer, in fondo, non è altro che una forma di demenza, che prende il nome dal neurologo tedesco, che nel 1907 fu il primo a descriverne le caratteristiche. Con il passare del tempo, le lacune mentali provocate da questa malattia diventano sempre più gravi, fino ad avere un'interferenza con le attività quotidiane. Almeno il 20 per cento dei casi di demenza vengono classificati come morbo di Alzheimer. A differenza del pensiero comune, l'Alzheimer non colpisce soltanto i pazienti in età molto avanzata, ma può insorgere anche prima dei Il periodo peggiore per la gestione di un paziente con l'Alzheimer va dalla manifestazione dei sintomi fino agli otto o dieci anni successivi, in cui la malattia progredisce inesorabilmente. L'unica cosa che al momento si può fare è dare supporto e sostegno sia ai familiari che ai pazienti. Ecco quindi il perché di campagne di sensibilizzazione nazionali che avvengono in questa giornata nelle circa 60 residenze, soprattutto per dare risalto ad un ruolo importante, quello dei *caregiver*. *(Applausi dall'interrogativo che dà nome alla campagna («E se le persone che ami sparissero?») e che richiama l'attenzione sugli effetti devastanti della malattia, le diverse iniziative di comunicazione enfatizzeranno l'importanza dell'affetto dei familiari. Quindi è qui che è importante l'affiancamento pratico ed emotivo dei malati, sia da parte dei familiari che dei *caregiver*, che sono molto importanti. Soprattutto, è importante trattare con amore una persona che ti urla in faccia, che non ti riconosce, che non sta ferma oppure che resta ferma con lo sguardo lucido nel vuoto e che non è più la buona o brava mamma o babbo, nonna o nonno, moglie o marito. E tutto questo per anni, sapendo che si può solo peggiorare, restare così per altri mesi, per poi peggiorare ancora. Ecco che allora si alternano momenti di sollievo con momenti di senso di colpa, quando si lasciano in custodia ad altri in residenze sanitarie. Ecco, io in questa giornata vorrei ricordare a tutti noi l'importanza di portare avanti un disegno di legge per il riconoscimento della figura dei *caregiver*, presentato dalla qui presente senatrice Bignami e firmato da ben 94 senatori, tra cui il sottoscritto. In questo giorno pensiamo anche a questa cosa. grazie a tutta